è particolarmente attento all'esigenza di agevolare l'ingresso in Italia di imprenditori e investitori provenienti da Paesi i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo di visto. A tal fine, negli ultimi anni sono stati adottate significative misure, volte a semplificare le procedure di richiesta di visto da parte di tali categorie di soggetti. In primo luogo, la Farnesina ha fissato in due giorni lavorativi il tempo d'attesa per l'emissione dei visti per affari. Si tratta della tipologia di visto d'ingresso utilizzata dagli uomini d'affari per soggiorni di breve periodo, fino a un massimo di novanta giorni, in area Schengen. Il visto per affari deve infatti essere emesso in tempi rapidi, per consentire agli operatori economici di recarsi nel nostro Paese anche con scarso preavviso, al fine di condurre trattative e partecipare a incontri con interlocutori attivi in Italia. Da una ricognizione dei dati in possesso dell'amministrazione risulta che la gran parte dei visti per affari venga effettivamente emessa entro due giorni dal momento della presentazione della domanda. A livello procedurale, i visti per affari seguono un *iter* semplificato, grazie allo strumento delle cosiddette liste bianche, adottate nella prassi dalle rappresentanze all'estero. Gli uffici commerciali dell'ambasciata *in loco* predispongono e aggiornano costantemente l'elenco delle imprese e degli imprenditori dei Paesi che hanno rilevanti rapporti economico-commerciali con il sistema Italia. Tale lista è condivisa con il corrispondente ufficio visti della rappresentanza diplomatica, il quale tratta le domande dei diretti interessati in via prioritaria, semplificando al massimo la relativa procedura e contenendo i tempi di trattazione delle istanze. Inoltre, per gli investitori che intendano trasferirsi stabilmente in Italia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri hanno recentemente introdotto un'apposita tipologia di visto, denominata Investor Visa for Italy. Le domande di visto per gli investitori vengono presentate e trattate attraverso un'apposita piattaforma informatica, che semplifica il processo di trattazione delle pratiche. Per stabilirsi in Italia, gli imprenditori stranieri hanno anche a disposizione altre tipologie di ingressi, quali lavoro autonomo e *startup*, che godono di canali prioritari presso gli uffici visti sul piano amministrativo e procedurale. In considerazione della struttura, dell'estensione della rete diplomatico-consolare e della varietà di tipologie di visto, la valutazione caso per caso a livello periferico delle esigenze della comunità imprenditoriale straniera consente di tenere in debito conto la peculiarità del contesto ambientale di riferimento e le costanti modifiche delle condizioni locali. In tal senso, il modello delle liste bianche consente un aggiornamento rapido e flessibile dell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni e di graduarle in base alle esigenze del singolo richiedente.

ringrazio il Sottosegretario per la sua risposta alla mia interrogazione che ritengo di fondamentale importanza trovando soddisfazione rispetto a quanto ha detto. In particolare, la richiesta di un visto per chi proviene da Paesi *extra* UE disagiati spesso è problematica. La necessità di investitori e imprenditori esteri che vogliono venire nel nostro Paese è quella di avere la possibilità di procedure di visto snelle che permettano di programmare la propria attività commerciale in tempi relativamente rapidi, e su questo lei mi ha dato soddisfazione. Molti investitori si trovano in grande difficoltà a partecipare a eventi fieristici e ad appuntamenti di lavoro non avendo certezza sui tempi di rilascio del visto. Sono molte le associazioni e le aziende italiane interessate all'argomento che ho avuto modo di incontrare in questi mesi, tra le quali Confindustria Ceramica e FederlegnoArredo, solo per citarne due. Tutti avrebbero beneficio nell'apertura di canali preferenziali per chi viene in Italia ad acquistare prodotti. Accolgo quindi con favore l'apertura del Ministero all'istituzione di queste procedure agevolate per chi voglia venire ad investire in Italia provenendo da Paesi *extra* UE, anche disagiati. Dal Continente africano, dal Sud Est asiatico, provengono quotidianamente richieste di visti di persone che sono interessate a visitare il nostro Paese per acquistare beni e macchinari e per partecipare a fiere di settore. Questa possibilità va senz'altro supportata. La *ratio* dell'istituzione di questo elenco va ricercata nell'importanza che gli investimenti esteri assumono sempre di più ogni anno per il *made in Italy*. Gran parte dei settori industriali e produttivi beneficiano di una crescita alla voce *export* e credo che agevolare le procedure per l'ottenimento dei visti di ingresso in UE sia un elemento imprescindibile per non correre il rischio della fuga verso altri Paesi. Ricordo che per l'ottenimento dei visti in Paesi come la Germania sono necessari pochi giorni (anche noi, come già detto, adotteremo presto queste procedure) e che potenziali investitori, di fronte alle difficoltà di ottenimento del visto in Italia, farebbero presto a rivolgersi altrove. Non sottovalutiamo anche in altri ambiti gli ostacoli della burocrazia; sono questi che da anni frenano la ripartenza della nostra economia.

Signor Presidente, stimati senatori, innanzitutto desidero ringraziare il senatore interrogante, poiché con il suo atto ispettivo mi consente di illustrare, anche in quest'Aula, le iniziative - alcune delle quali di natura legislativa

eppure, nonostante le numerose sollecitazioni manifestate nella scorsa legislatura anche in sede parlamentare, nulla di concreto è stato fatto finora per garantire una tutela qualificata e differenziata

I fattori di rischio responsabili di tali atti di violenza sono numerosi, ma l'elemento peculiare e ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga. Ecco perché si ritiene che il Servizio sanitario nazionale, a differenza di altri ambiti, abbia una doppia responsabilità: quella di prendersi cura e tutelare i soggetti che necessitano di cure, nonché quella di tutelare la sicurezza e il benessere fisico del personale sanitario che vi opera. Gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari sono peraltro considerati eventi sentinella, in quanto rappresentano segnali della presenza nell'ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità, che richiedono l'adozione di opportune misure di protezione dei lavoratori. A fronte di questa consapevolezza, il Ministero della salute ritiene di dover intervenire attraverso una pluralità di misure che possano consentire - viste nel loro insieme, in un'ottica di sistema - la realizzazione di risultati concreti e, soprattutto, duraturi. Prima di tutto, si impone, come appena detto, un approccio preventivo che consenta di conferire sicurezza, sotto tutti i punti di vista, all'ambiente di lavoro degli operatori sanitari. In coerenza con tale impostazione, che riconosce importanza anche alle condizioni quotidiane di lavoro degli operatori sanitari, il 3 luglio scorso, il Ministero della salute ha istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel cui ambito si intende rivolgere una particolare attenzione ai fenomeni, purtroppo sempre più frequenti anche in sanità, delle aggressioni al personale medico e non medico. Sempre nella accennata ottica preventiva, ricordo che proprio quest'Assemblea ha appena approvato il decreto-legge sicurezza e immigrazione, al cui interno si è voluta inserire una specifica disposizione che rafforza la tutela preventiva dei presidi sanitari. Mi riferisco all'estensione del Daspo urbano introdotto dal cosiddetto decreto Minniti, anche ai presidi sanitari. Approfitto, anzi, di questa occasione per chiarire meglio i contorni di questo istituto che qualcuno ha voluto erroneamente nominare Daspo sanitario, evidentemente senza comprenderne bene il contenuto. Il decreto Minniti - con disposizioni che non sono state ritoccate, per quanto qui di interesse - ha concesso una mera facoltà ai sindaci di individuare, nell'ambito del proprio territorio, quei luoghi pubblici da tutelare, sotto il profilo del decoro urbano, attraverso l'introduzione di una sanzione pecuniaria e di un obbligo di allontanamento a carico dei soggetti che, con il loro comportamento, ne impediscano l'accesso o la fruizione ad altri. La concreta individuazione di tali siti era - ed è ancora - rimessa ai sindaci che possono rintracciarli nell'ambito di una più ampia tipologia di luoghi pubblici già fissata dal decreto Minniti (scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibiti a verde pubblico) ai quali, con il recente decreto sicurezza, si sono dunque aggiunti anche i presidi sanitari (oltre che le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli). Si tratta, con tutta evidenza, di misure assolutamente preventive, oltre che proporzionate e differenziate, in quanto calate sui territori a seguito di scelte effettuate dal livello di governo di maggiore prossimità, quale è il Comune. Misure che, in definitiva, lungi dall'impedire la fruizione delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, magari anche i più bisognosi - circostanza, questa, mai posta in discussione - serviranno, in un'ottica preventiva, a disincentivare comportamenti non consoni, agevolando, e non ostacolando, l'accesso ai presidi sanitari, in un contesto di maggiore sicurezza di cui beneficeranno, ovviamente, anche gli stessi operatori sanitari. L'altra importante iniziativa già avviata da questo Governo riguarda, come ormai noto, lo specifico disegno di legge - che inizierà il proprio *iter* da questo ramo del Parlamento - che si è voluto dedicare al fenomeno della violenza sugli operatori sanitari. Da una parte, considerato che il Ministero della salute non dispone di dati certi di tutti gli episodi di violenza a danno degli operatori nel territorio nazionale, e nella consapevolezza di dover affrontare il fenomeno anche attraverso un attento monitoraggio degli episodi stessi, nel disegno di legge si propone la costituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il personale della sanità, con la presenza di rappresentanti delle Regioni e dei Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro. L'osservatorio ha il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di promuovere studi ed analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori

Dall'altra parte è stata prevista quale specifica aggravante di pena l'aver commesso atti di violenza e minacce nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni: una misura che conferisce un regime di tutela particolarmente rafforzato agli operatori sanitari, certamente in grado di accrescere la deterrenza dalla commissione dei predetti reati. Concludo, dunque, confidando che il Parlamento voglia accogliere con favore queste proposte normative che vanno nella direzione (che - mi permetto di dire - non può conoscere divisioni politiche) della maggiore tutela della dignità del lavoro di tutti gli operatori sanitari.

fare un'osservazione in premessa rispetto alla risposta che lei, signor Sottosegretario, mi ha dato. Noi non possiamo trattare questo tema esclusivamente come una questione che ha a che fare con l'ordine pubblico, perché non è un caso che la stragrande maggioranza degli episodi di aggressione nei confronti del personale medico o della sicurezza in genere negli ospedali avviene nei luoghi dove gli ospedali funzionano meno.

si indicano in rosso i luoghi in cui tali episodi avvengono più frequentemente, si nota che il Mezzogiorno è quasi il luogo esclusivo dove si verificano fenomeni di aggressione nei confronti del personale medico. Questo è direttamente collegato a come funziona il nostro sistema sanitario. Nulla può giustificare un'aggressione, per cui va condannata e assolutamente colpita, fare un ragionamento su come far funzionare meglio le nostre strutture ospedaliere, e quindi su come ridurre anche un fenomeno che alimenta ed incentiva le condizioni di disordine pubblico negli ospedali, sicuramente è importante. Pertanto, quello che io chiedo al Governo - ed era il motivo della mia interrogazione è di intervenire in maniera più incisiva nei confronti delle Regioni sui temi che riguardano pronto soccorso, liste d'attesa e funzionamento delle strutture. Ciò va fatto soprattutto da parte di chi ha

più sicurezza, più attenzione, più sostegno alle Forze dell'ordine e al personale medico in ospedale, ma al tempo stesso bisogna agire per far funzionare meglio gli ospedali, come strumento migliore per ridurre i disordini nelle strutture sanitarie.

Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la disciplina di arruolamento della categoria dei lavoratori marittimi, rappresento quanto segue. Come riportato dagli onorevoli interpellanti e già specificato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 24 del 2014, la richiamata disciplina in materia di contratto a termine contenuta nel codice della navigazione risulta di carattere speciale. L'articolo 1 del codice prevede infatti che: «In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano le disposizioni presenti all'interno del codice nonché le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi». La stessa disposizione prosegue stabilendo che: «Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile». Per quanto riguarda la disciplina in materia di contratti a termine per il personale navigante, dunque, bisogna fare riferimento espressamente al codice della navigazione, che essendo norma speciale deroga alla normativa ordinaria in materia. In particolare, l'articolo 325 stabilisce che: «Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato». Inoltre: «Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro». In particolare: «La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita: a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio; b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo; c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito; parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti». Il successivo articolo 326, peraltro riportato dagli onorevoli interpellanti, stabilisce invece che: «Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; ogni stipula di durata superiore, si considera a tempo indeterminato.». Inoltre: «Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato». Agli effetti di ciò che è previsto nell'articolo 326, come espressamente indicato al comma successivo: «La prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta In relazione a quanto esposto nell'interrogazione, e alla luce di quanto espressamente indicato all'interno della normativa, evidenzio, come indicato nell'interpello n 24 del 2014 del Ministero del lavoro che in merito alla successione delle suddette tipologie di lavoro a termine, la norma in questione - considerando altresì ininterrotta la prestazione resa nelle ipotesi in cui tra un contratto e l'altro non intercorra un periodo superiore a sessanta giorni - appresta delle tutele avverso eventuali abusi rispetto all'utilizzo di tale forma contrattuale. A ogni buon conto, rappresento che, nell'ambito del prossimo documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2019, da adottarsi in sede di commissione centrale presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3 del decreto legislativo n. 124 si darà specifico risalto alla necessità di verificare il rispetto della disciplina sui contratti a tempo determinato. Infine, questo Dicastero - attraverso un coordinamento con i colleghi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per materia sul codice della navigazione - avvierà un'approfondita valutazione della problematica descritta dagli onorevoli interpellanti, al fine di scongiurare il reiterarsi delle pratiche in uso nel settore dei lavoratori marittimi. Come già fatto con l'approvazione del decreto dignità, questo Governo ha come obiettivo fondamentale la dignità dei lavoratori attraverso la riduzione del precariato e l'aumento delle tutele di tutte quelle categorie di lavoratori maggiormente esposti.

signor Sottosegretario, la ringrazio per la lunga e articolata risposta. Mi ritengo soddisfatto. Il Governo ha toccato i due temi fondamentali: i controlli e la precarizzazione del lavoro. Sono molto preoccupato, però, per la situazione del comparto. È veramente insostenibile. Lo sappiamo, la questione dei marittimi nasce nel 1998, quando le nuove norme consentirono l'imbarco a prezzi stracciati di personale non italiano che doveva favorire gli armatori e che, invece, ha messo in ginocchio la marineria italiana. Mentre i ragazzi italiani escono dagli istituti nautici e non trovano lavoro né possibilità di formarsi e fare carriera nella marina mercantile, gli armatori, con il tacito consenso della politica, hanno imbarcato sempre più personale straniero o extracomunitario, inferiore di tre o quattro volte quelli italiani, sui quali gli armatori hanno continuato a usufruire delle agevolazioni, anche a causa dei mancati controlli e, soprattutto, a causa di un totale disinteresse della politica stessa. La nostra è una delle marinerie più esperte al mondo e in questi anni - come ha ricordato anche il ministro Di Maio - è stata vittima dei *business* più disparati, da quello della formazione (una volta pubblica e oggi a pagamento) a quello delle assunzioni. I risultati di queste politiche scellerate sono stati migliaia di marittimi italiani disoccupati, equipaggi sottopagati e - terzo, ma non ultimo - il progressivo smantellamento dell'ennesimo comparto strategico per la nostra Nazione. Sono convinto che, grazie a questo Governo del cambiamento, finalmente le norme saranno applicate e i benefici fiscali del registro internazionale saranno limitati alle navi che imbarcano solo equipaggi italiani o comunitari sulle rotte di cabotaggio e di continuità. Il mondo va verso la progressiva riduzione del personale imbarcato sulle navi e a minore quantità di personale corrisponderà una sempre maggiore richiesta di professionalità e specializzazione. La nostra marineria e i nostri marinai sono in grado di essere ai vertici mondiali e per questo devono essere valorizzati e non sfruttati, sottopagati o sottoccupati. Una legge entrata in vigore questa estate avrebbe risolto molti dei problemi indicati, ma tre anni dalla sua approvazione non sono bastati per renderla operativa, né si sa quando potrà dispiegare i suoi effetti. Sono convinto che il nostro Governo avrà la sensibilità, l'intelligenza e la lungimiranza di risolvere questa annosa questione. Il nostro Paese ha bisogno di questo settore e ha bisogno dei nostri marittimi. Difendiamoci e difendiamoli.

sono avvenute vicende che in questo momento rendono urgente porre al Governo domande leggermente diverse da quelle contenute nell'interpellanza. La Bekaert è un'azienda molto importante della Toscana centrale. Si trova nel Valdarno, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e occupa 318 lavoratori. è stata oggetto, qualche anno fa, di un'acquisizione da parte di una multinazionale con sede in Belgio, che nei mesi scorsi ha annunciato la volontà di chiudere lo stabilimento, in una maniera che ha suscitato sconcerto nel Governo stesso, che ha visitato lo stabilimento con il Ministro per lo sviluppo economico, in tutta la comunità locale, tra i cittadini e nelle istituzioni locali, come la Regione e l'amministrazione comunale. C'è stata una diffusa solidarietà e in molti si sono pronunciati per scongiurare l'azione predatoria annunciata dalla Bekaert. In questo momento siamo in una situazione caratterizzata dal ripristino della cassa integrazione straordinaria per cessazione,

C'è però un problema che resta aperto, perché ovviamente il ripristino della cassa integrazione per cessazione crea un'opportunità ma non può rappresentare un un modo di risolvere il problema. La soluzione del problema è soltanto nella reindustrializzazione, quindi nella ricerca di un investitore serio che dia nuova vita a questo stabilimento, nello stesso settore in cui oggi opera o in un altro. Quello che io chiedo al Governo è di specificare che cosa si sta facendo affinché la ricerca di questo investitore dia frutti. Sappiamo bene, per aver visto tante vertenze di questo tipo, che è importante trovare non un investitore qualsiasi ma soggetti dotati di serietà, che siano qualificati e che non ripropongano modi di agire che così tanta preoccupazione, e poi alla fine anche danni, hanno creato in questo territorio. Bisogna che questa ricerca sia incalzante e intensa; il Ministro dello sviluppo economico e la sua squadra possono e devono svolgere un ruolo molto importante e incisivo. Credo sia inoltre importante che vengano tenuti costantemente informati degli sviluppi che ci sono le comunità e le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e i lavoratori, che ovviamente si trovano in una condizione di angoscia che la reintroduzione degli ammortizzatori sociali ha solo attenuato ma non può cancellare. Come Partito Democratico, attraverso i nostri europarlamentari, abbiamo anche avuto un incontro, il 12 settembre, con il commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, per capire se c'erano state violazioni delle regole europee nelle scelte della multinazionale belga Bekaert. È stata aperta un'istruttoria e, per il momento, non paiono esserci violazioni. Del resto a questa vicenda - vorrei chiarirlo - non si può applicare nemmeno la clausola antidelocalizzazioni che è stata introdotta in uno dei provvedimenti varati prima della pausa estiva dal Governo, perché si tratta di un'azienda che ha sede nell'Unione europea e che vuole delocalizzare la produzione figlinese in un altro paese dell'Unione europea, segnatamente la Romania. Noi abbiamo condiviso la scelta della reintroduzione della CIGS per cessazione. Tra l'altro, ciò è stato fatto con i fondi stanziati dalla riforma del lavoro del 2015 e importando letteralmente la causale che quella riforma prevedeva per le ristrutturazioni. Però ovviamente abbiamo grande preoccupazione in merito alla possibilità di trovare in tempi brevi una soluzione di reindustrializzazione. Chiediamo al Governo il massimo impegno e chiediamo anche se ci sono notizie, perché ovviamente tutta una comunità, quella che si è schierata in difesa dei lavoratori, attende con il fiato sospeso che ci siano evoluzioni positive.

l'onorevole interrogante ha già dato sostanzialmente la risposta, che comunque ovviamente completo con le informazioni che ho raccolto. Il Ministero dello sviluppo economico segue, dal 2016, gli avvenimenti della multinazionale belga Bekaert.

le attività lavorative per 318 dipendenti, per delocalizzare in Romania, senza alcun preventivo confronto e senza alcuna spiegazione sulle vere ragioni che hanno indotto la proprietà ad un atto così grave. Tale decisione ha destato notevoli perplessità, in quanto in un precedente incontro svoltosi al Ministero dello sviluppo economico il 29 marzo 2018 i rappresentanti della multinazionale in questione avevano illustrato un piano concernente gli obiettivi e l'avanzamento dei propri progetti in corso relativi al sito di Figline Valdarno, affermando che la *mission* dello stabilimento era quella di diventare *leader* nel settore dell'industrializzazione dei rinforzi d'acciaio per pneumatici. In tale sede, inoltre, veniva prospettato, alla luce di un forte peggioramento dei risultati aziendali, l'impegno a discutere comunque con le organizzazioni sindacali percorsi e soluzioni condivise con i lavoratori. Il 27 giugno 2018, in un'ulteriore riunione alla quale parteciparono i rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali, nonché le organizzazioni sindacali, ma non i rappresentanti della Bekaert, il Ministero dello sviluppo economico ha ribadito sia la gravità della decisione in sé, considerata dannosa per le famiglie coinvolte e l'economia del territorio, sia i modi in cui la stessa fu presa, posto che era stata adottata senza alcuna forma di contraddittorio, a differenza di quanto era stato in precedenza dichiarato. Il Ministero dello sviluppo economico, di conseguenza, ha chiesto con forza la revoca immediata dei licenziamenti e l'avvio di un confronto più serio e concreto. In data 30 luglio 2018, in un ulteriore incontro, si è data lettura di un piano prospettato e inviato dalla Bekaert al Ministero dello sviluppo economico per risolvere le problematiche che sarebbero derivate dalla chiusura del citato sito. Tale piano, tuttavia, nonostante evidenziasse una maggiore disponibilità da parte della proprietà, non soddisfaceva la principale richiesta manifestata dalle organizzazioni sindacali, ossia la sospensione della procedura di mobilità collettiva. Finalmente, dopo molteplici contatti, interlocuzioni e incontri, il 3 ottobre scorso, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, è stato siglato un accordo sul piano sociale e sui nuovi ammortizzatori per i lavoratori dello stabilimento di Figline Valdarno della multinazionale belga Bekaert. Con tale accordo sono stati previsti una pluralità di strumenti, incentivi e attività finalizzati alla reindustrializzazione del sito e al ricollocamento dei lavoratori, nonché una serie di misure - mi fa piacere ribadirlo - a tutela di questi ultimi. Tra queste, voglio ricordare la sospensione della procedura di licenziamento collettivo; la cassa integrazione della durata di un anno, a partire dal 1° gennaio 2019 (possibilità resa possibile dall'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109); incentivi all'esodo, che prevedono tre scaglioni di anzianità per ogni fascia. Nello stesso è anche riscontrabile l'impegno dei vari soggetti presenti sul territorio - dalle imprese alle istituzioni locali - che hanno condiviso l'obiettivo di voler recuperare la crisi della Bekaer, incentivando, da un lato, i nuovi soggetti che potrebbero essere interessati a insediarsi in quell'area produttiva e, dall'altro, premiando chi deciderà di assumere i lavoratori altrove. In relazione al piano industriale, mi preme sottolineare che la produzione dell'azienda continuerà fino al 31 dicembre 2018 e la sua attuazione sarà monitorata dal Ministero dello sviluppo economico attraverso incontri con le parti a cadenza mensile. Tali fatti dimostrano che il Ministero dello sviluppo economico ha posto la massima attenzione sulla vicenda Bekaert e si è attivato e concretamente impegnato per trovare una soluzione alle problematiche connesse. In particolare lo stesso ha agito in via generale attraverso una stretta al fenomeno delle continue delocalizzazioni che affliggono il Paese, con l'introduzione di sanzioni alle imprese che

che l'introduzione della cassa integrazione per cessazione dà una boccata di ossigeno ma non rappresenta una soluzione. L'accordo che è stato stipulato il 3 ottobre evita il precipitare delle cose, ma, di per sé, non rappresenta la garanzia che, alla fine dell'anno di cassa integrazione, di dare un futuro industriale a questo stabilimento e lavoro ai lavoratori colpiti dalla scelta della Bekaert. Mi pare di capire che le attività finalizzate all'individuazione di un investitore serio e qualificato, che possa rilevare lo stabilimento e farlo oggetto di una reindustrializzazione, sono in una fase preliminare e non ci sono ancora sbocchi concreti sul campo. Raccomando allora la massima attenzione; il ruolo che potrà e vorrà svolgere il Ministero per lo sviluppo economico è essenziale perché sappiamo bene che le reindustrializzazioni non piovono dal cielo,

il problema le comunità locali, i sindaci e tutte le forze che sono in grado di sollecitare interessi di impresa che possano tradursi nella soluzione del problema. Rinnovo anche la richiesta di di tenere costantemente informati lavoratori, organizzazioni sindacali, il sindaco del Comune dove lo stabilimento ha sede e tutte le forze locali, degli sviluppi che ci sono, perché avere tutti un'informazione aggiornata ed essere tutti allineati sul piano delle informazioni consente di fare meglio il lavoro di squadra che i lavoratori ci chiedono. Del resto siamo di fronte ad una vicenda in cui i colori politici devono fare un passo indietro e tutti dobbiamo spingere perché si possa superare un problema che ha generato angoscia e preoccupazione molto forti in un'intera comunità.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'interno, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per la pubblica amministrazione.

colleghi, negli ultimi anni sia il Ministero dell'interno che il Ministero degli affari esteri hanno provveduto a introdurre semplificazioni burocratiche finalizzate a snellire le procedure di rilascio del passaporto. In particolare, qualche anno fa, proprio il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha stipulato una convenzione con Posteitaliane SpA per l'attivazione di un servizio per la consegna a domicilio del documento. Nonostante le semplificazioni introdotte sul lato delle autorizzazioni e del ritiro del passaporto, sono rimaste però invariate tutte le altre incombenze preliminari. Per questo motivo, il cittadino è ancora obbligato a presentare un contrassegno telematico (da euro) che deve acquistare in una rivendita di valori bollati e la ricevuta del versamento di 42,50 euro, da effettuarsi esclusivamente presso gli uffici postali. Si tratta di adempimenti che, a prescindere dai costi sostenuti, costituiscono ancora un appesantimento burocratico relativamente ai tempi complessivi dell'intera procedura, il tutto a svantaggio del cittadino. Da anni, l'intera attività amministrativa pubblica è incentrata sulla messa in atto di un processo di sburocratizzazione generale che, sulla base dei criteri di economicità e di efficacia, snellisca i procedimenti, favorendo la digitalizzazione e semplificando il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i privati. Per questi motivi, le chiedo, signor Ministro, se lei non ritenga ipotizzabile l'introduzione di ulteriori semplificazioni, finalizzate a snellire anche le incombenze preliminari, ad esempio prevedendo uno sportello unico presso il quale

imprese, pratiche edilizie. È priorità della Lega e dell'intero Governo rendere più semplice la vita ai cittadini, andando meno in giro presso vari sportelli e compilando meno moduli. Tornando al tema cui lei si riferisce, il Ministero dell'interno ha stipulato nell'ottobre del 2014 una convenzione con Posteitaliane SpA per offrire ai cittadini, appunto per snellire gli oneri burocratici, la possibilità di ricevere al proprio domicilio il passaporto elettronico. Tale convenzione scade il 31 dicembre di quest'anno ed è attualmente in fase di rinnovo. Noi stiamo lavorando per migliorare questa convenzione. Al fine di facilitare ulteriormente la procedura di rilascio del documento di viaggio dal pagamento degli oneri economici, quali il contrassegno amministrativo e il versamento per il rilascio del documento, è attualmente allo studio - e ci stanno lavorando i miei uffici - un'ipotesi di fattibilità per la semplificazione delle citate procedure attraverso un sistema di pagamento elettronico unificato. In particolare se ne sta valutando la possibile applicazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, che consente i pagamenti verso la pubblica amministrazione in modalità informatica standardizzata, attraverso i prestatori di servizi di L'obiettivo è ovviamente rendere tali pagamenti effettuabili direttamente dal cittadino sul portale o sulla *app* dell'ente, ovvero attraverso i canali di interconnessione di banche o altri sportelli, quali le agenzie, l'*home banking*, gli sportelli ATM o gli uffici postali. Tale ipotesi vede peraltro il favore del Ministero degli affari esteri e ci sta lavorando la collega Bongiorno per quanto riguarda la funzione pubblica. Lo stesso Ministero degli affari esteri ha già attivato tale modalità semplificata di richiesta del passaporto per i cittadini italiani residenti all'estero, che possono effettuare, in una unica soluzione, senza fare il giro delle diciotto chiese, il pagamento della commissione amministrativa e del costo del libretto direttamente all'ufficio consolare in valuta locale. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. *(Applausi dai

Non siamo fanalino di coda, perché l'Italia ha su questo fronte un primato non da conquistare, ma da mantenere. Quindi spero che, al più presto, il Governo riesca a ottenere anche questa semplificazione,

*(M5S)*. Signor Ministro, nella legge di bilancio per il 2018 sono state inserite, tra le altre, alcune norme in materia di stabilizzazione per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nel particolare, si tratta di una riserva di posti, nell'ambito di procedure straordinarie di assunzione, per i cosiddetti precari discontinui iscritti nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo, in possesso di determinati requisiti. A norma del decreto legislativo n. 139 del 2006 tale personale, infatti, può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Come ben ricorderà, signor Ministro, il tema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro è presente anche all'interno del contratto di Governo. Mi fa piacere notare che anche nella legge di bilancio per il 2019, all'articolo 31, comma 3, sono già previste assunzioni anche per questo personale, seppure in subordine. Questo fatto dimostra che l'attenzione del Governo è comunque alta sulla materia. Dobbiamo ricordare come nel caso di eventi meteorologici straordinari - e purtroppo in Italia sono fenomeni sempre più frequenti - gli interventi in coda per le richieste di aiuto ai Vigili del fuoco siano spesso piuttosto numerose. Per questo è importante dare seguito alle previsioni legislative e assicurare la stabilizzazione del rapporto di lavoro di personale che è già formato e in grado, *in primis*, per la sicurezza dei cittadini, di assicurare interventi tempestivi e adeguati *standard* di efficienza. Quindi, signor Ministro, le chiedo quali misure siano state intraprese e quali si intendano intraprendere, comprese tempistiche e modalità operative, per ottemperare alle disposizioni che prevedono l'assunzione di tali contingenti di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i cosiddetti precari discontinui, e quali iniziative

Grazie senatrice Granato, penso che l'Assemblea del Senato potrebbe approfittare della diretta televisiva per tributare a questi eroi, che sono i Vigili del fuoco, l'applauso per quello che fanno quotidianamente al servizio della nostra comunità.

Venendo al tema dell'interrogazione, intendo sottolineare come il Ministro dell'interno abbia da sempre avvertito l'esigenza di valorizzare - da ben prima di me, evidentemente - e non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario dei Vigili del fuoco a sostegno della capacità operativa dell'intero apparato del soccorso tecnico urgente. Diverse sono state le iniziative, anche di carattere normativo, in tal senso: mi riferisco alle recenti disposizioni che hanno elevato dal 25 al 35 per cento la riserva di posti in favore dei volontari nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione della qualifica di vigile del fuoco e a quelle che hanno introdotto un'ulteriore riserva del 10 per cento dei posti disponibili in tutti gli altri concorsi di accesso nei ruoli del Corpo nazionale. Alla stabilizzazione dei volontari sono dedicate anche le misure - richiamate contenute nella legge di bilancio dell'anno scorso, quindi del 2018, con le quali si prevede un'assunzione straordinaria di vigili del fuoco, riservata al personale volontario, nel limite del 30 per cento dei contingenti annuali. Questo ci consentirà, nell'arco di un quinquennio, di stabilizzare 480 volontari in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ulteriori 28 unità di personale volontario, con particolare riferimento ai nuclei cinofili

Al fine di avviare le predette procedure di stabilizzazione, informo che lo scorso 26 ottobre - quindi dieci giorni fa - ho firmato il decreto che individua le modalità abbreviate del corso di formazione, i criteri di verifica dell'idoneità operativa del personale discontinuo e le modalità di espletamento delle procedure Inoltre, nel decreto sicurezza, la cui conversione quest'Assemblea ha approvato ieri, sono stati incrementati gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco di 6 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro a partire dal 2020, aumentando i richiami annui.

abbiamo previsto l'assunzione di 1.500 vigili del fuoco secondo la seguente tempistica: 650 uomini dal 10 maggio 2019; 200 dal 1º settembre 2019; altri 650 dal 1º aprile 2020. 2020. In occasione di tale potenziamento dell'organico, sarà possibile procedere alla stabilizzazione di ulteriori 195 volontari discontinui. Mi sembra che numeri, cifre e date

sacrifici personali anche ingenti, per mantenersi sempre addestrati e preparati, costi

concreti, che chiaramente ci stanno a cuore. La interrogo, quindi, signor Ministro, sul tema del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Premetto, però, prima di entrare brevemente nel merito, che chi vi parla è un cattolico liberale, non un oscurantista ma un fervido democratico, una persona che, però, come tutti noi della destra italiana, sente particolarmente, nel proprio cuore e nel proprio pensiero, il rispetto dell'etica e dei propri Ebbene, signor Ministro, in questi ultimi mesi anche nel mio Trentino sono avvenuti casi di iscrizione negli atti dell'anagrafe di figli nati secondo tecnicalità che costituiscono reato nel nostro Paese. Parlo di utero in affitto e di fecondazione eterologa, cioè di tecnicalità che non sono permesse a coppie

e magari inficiata da una cultura libertaria che tutto ha permesso. Ciò ha portato, quindi, ad ottenere il riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso. A questo punto, io le chiedo,

Soprattutto, che non si giochi sulla pelle dei figli, perché le abitudini sessuali di ciascuno sono tutelate da chiunque, e ne sono io il primo sostenitore, ma la crescita dei figli deve avvenire anche secondo il rispetto dei nostri valori, della nostra tradizione.

premetto che rispondo a un atto che è prevalentemente inerente a una materia, quella dello stato civile, per la quale è competente il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 54 del testo unico degli enti locali. Al riguardo, sentiti i competenti uffici del predetto Ministero, rappresento quanto segue. Le vicende relative alle modalità di iscrizione e trascrizione di atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali costituiscono oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali. Tra i numerosi esempi che potrebbero essere evocati al riguardo, mi limito a richiamare i casi, emersi di recente, di richieste di trascrizioni integrali dell'atto di nascita estero indicante due madri, ovvero due padri, di richieste di iscrizione nell'apposito registro dell'atto di nascita italiano indicante due genitori dello stesso sesso e di richiesta di trascrizione della sentenza straniera che modifica l'atto di nascita estero, indicante un solo genitore, così già trascritto in Italia, mediante l'aggiunta di un secondo genitore dello stesso sesso. Nel merito della questione, posso anzitutto ribadire quanto affermato in precedenza dal Ministro dell'interno in risposta ad analogo atto di sindacato ispettivo, ossia che esistono alcuni punti fermi. Il primo è che secondo il vigente ordinamento di stato civile gli atti di nascita si formano e si iscrivono nei relativi registri indicando, quali genitori, la madre partoriente ed il padre biologico. Tale principio viene anche riaffermato con riferimento all'annotazione nell'atto di nascita del riconoscimento di filiazione che richiede, sempre, la preventiva verifica in capo al soggetto dichiarante della condizione di paternità o di maternità. Il secondo è che l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, ha considerato le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani quali fattispecie delittuose. D'altro canto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 272 del 2017, ha sottolineato che «la maternità surrogata è una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Dunque, se il divieto di gestazione per altri è presente nel nostro ordinamento va fatto rispettare in termini concreti, evitando che il ricorso all'estero a tali pratiche si traduca, poi, con l'ingresso in Italia del minore in un continuo aggiramento di un divieto che nell'ordinamento nazionale è volto a preservare valori fondamentali, quali, innanzitutto, la dignità della donna, che rischia in questo modo di essere ridotta a mero oggetto.

che vengano iscritti figli a genitori dello stesso sesso. A questo proposito, mi permetto anche di ricordare al signor Ministro e al Governo che il Gruppo Fratelli d'Italia, mio tramite come primo firmatario e con la collega Rauti come secondo firmatario, ha presentato in data 19 giugno, quindi ben cinque mesi fa, uno specifico disegno di legge, per normare in modo inequivocabile e collegare quindi il pensiero e la filosofia con la concretezza, come vorremmo. Invito dunque il signor Ministro e il Governo a fare in modo che tale disegno di legge venga al più presto incardinato e possa portare a una risposta chiara, che riguarda tutti noi, la vita e la crescita dei nostri figli.

Ministro, la sua forza politica, la Lega, ha proposto nella mia Regione il rilancio dei consultori e lei ha proposto anche il ripristino dei punti nascita chiusi nel nostro Paese e sgravi contributivi per le imprese che mantengono le madri al lavoro dopo la nascita dei figli.

le adozioni internazionali sono calate in questi anni e nella proposta che il suo Governo ha fatto in questi giorni ne propone rilancio. Le chiedo, dunque, anche a proposito di tale questione, in vista della legge di bilancio e dei prossimi provvedimenti, come intende procedere concretamente e fattivamente.

offerta, per iniziare un po' a parlare delle misure che il Governo intende adottare in favore della famiglia e che sono in parte già contenute nel disegno di legge di bilancio e in parte sono in corso di definizione per l'esito dell'esame parlamentare. In legge di bilancio siamo riusciti a ottenere, per la famiglia, 300 milioni di euro per il triennio 2019-2021 e ulteriori 100 milioni di euro per ogni anno successivo. Anticipo che intendo stanziare questi fondi prioritariamente per il *welfare* aziendale, per sostenere le aziende che fanno investimenti *pro* famiglia e *pro* natalità. A questo riguardo ho aperto anche un tavolo tecnico, nel quale si lavora sulle migliori esperienze già in atto. In bilancio è inoltre previsto, tra le altre cose, un incremento di 120 milioni di euro all'anno per le politiche sociali e di 100 milioni di euro - a regime - sul fondo per le non autosufficienze, che passa così da 450 milioni di euro l'anno Ricordo che il tema delle non autosufficienze e della presa in carico è strettamente connesso ai temi familiari. Riguardo alle misure per gli asili nido, saranno stanziati 960 milioni di euro nel prossimo triennio e stiamo lavorando per rendere la misura realmente efficace e fruibile, nonché per garantirne - laddove possibile - un incremento del 50 per cento. Possiamo, quindi, affermare che l'investimento complessivo in bilancio per la famiglia supera, ormai, il miliardo di euro. Ma ovviamente vogliamo fare ancora di più. A tutela della maternità, argomento a me molto caro, proporrò misure volte a garantire una maggiore flessibilità nella fruizione del congedo di maternità, sia con riguardo al limite di età del figlio entro il quale è possibile ottenere il congedo, sia con riguardo al trattamento economico percepito. In particolare, intendo innalzare fino a sedici anni - rispetto agli attuali dodici vigenti - l'età del figlio entro la quale al genitore è consentito di accedere al congedo; proporrò una flessibilità in contrazione e su base volontaria, concedendo alla madre che lo richiede la possibilità di usufruire di un congedo di tre mesi con indennità al 60 per cento della retribuzione, in alternativa agli attuali sei mesi al 30 per cento dello stipendio; prevederò, poi, ulteriori misure di conciliazione vita-lavoro come la facoltà di rendere ulteriormente flessibile il congedo di maternità; interverrò, inoltre, oltre che sulle misure relative alle assistenti materne, anche a favore della promozione del lavoro agile, dando priorità alle richieste di esecuzione di tale tipologia di lavoro alle lavoratrici nei tre anni successivi al periodo di fruizione del congedo di maternità, nonché a quelle con figli in situazione di disabilità. È in fase di approfondimento, per valutarne la compatibilità finanziaria dell'IVA a zero, o comunque agevolata per chi

ho soltanto due minuti, che sono per me sufficienti ad esprimere la mia disapprovazione e il mio sdegno per il suo silenzio rispetto alle parole di Rocco Casalino nei confronti delle persone Down, il mio sdegno e la mia disapprovazione per il suo silenzio nei confronti di Beppe Grillo quando ha attaccato, insultato, offeso le persone autistiche. Lei è lì e fa delle crociate per idee che non condivido sulla famiglia, però la vedo determinato. Al tempo stesso, non vedo le stesse crociate e la stessa determinazione nel difendere le persone con disabilità. Lo dico con dispiacere, perché credo che lei, quando ha assunto la carica di Ministro della disabilità, ha assunto il ruolo di una sorta di sindacalista delle persone disabili e delle loro famiglie. Oggi guardavo le agenzie con ansia con ansia cercando una sua dichiarazione che dicesse qualcosa nei confronti di uno che è portavoce del Presidente del Consiglio: non è un passante, ma il portavoce del Presidente del Consiglio, quindi è pagato dallo Stato; sta lì ed ha insultato le persone disabili e i ragazzi Down in particolare. Noi ci aspettiamo da lei una difesa. Non ci sono ragioni di partito, non ci sono ragioni legate alla necessità di tenere in piedi un Governo. Se qualcuno attacca le persone disabili, al di là di chi esso sia, lei ha il dovere, da Ministro della disabilità, di dire che quel qualcuno sta facendo una porcheria.

risulta che per il settore del pubblico impiego sono state stanziate nuove risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente delle prossime amministrazioni del triennio 2019-2021. Tali risorse, che vanno calcolate al netto delle entrate contributive e fiscali che generano, risultano pari a 700 milioni nel 2019, un miliardo nel 2020 e 1,3 miliardi a decorrere dal 2021, mentre per le assunzioni di personale del settore statale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sono stati stanziati 230 milioni nel 2019, 570 milioni nel 2020 e 760 milioni nel 2021.

per il reddito di cittadinanza, peraltro con la singolare iniziativa di stanziare risorse in *deficit*, cioè chiedendo soldi agli italiani, cioè ai nostri cittadini, attraverso l'emissione di nuovo debito pubblico. Questo è tutto ciò che si può trovare nella legge che destina risorse a vari comparti della pubblica amministrazione, in cui sono comprese anche le assunzioni per i fondamentali comparti delle Forze di polizia, che poco fa il ministro Salvini ricordava

noi servono da subito. Le chiedo, signor Ministro, se abbia davvero un piano preciso per affrontare in modo organico gli enormi problemi che derivano da una pubblica amministrazione spesso organizzata male,

infatti non si deve assumere personale per farlo stare dietro le scrivanie, ma in certi settori: digitalizzazione, semplificazione, uso dei fondi europei. Nel disegno di legge di bilancio abbiamo anche indicato le modalità attraverso le quali attuare il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento delle *performance*. Tuttavia, visto che lei faceva riferimento a dei numeri, è giusto che io le risponda con dei numeri. Nel disegno di legge di bilancio sono previste consistenti assunzioni che si aggiungono a quelle ordinarie, in relazione alle quali sono stati stanziati, per il triennio 2019-2021, complessivi 870 milioni di euro. Devo dire, ma già risultava dalla risposta del ministro Salvini, che credo sia innegabile l'attenzione ai settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, della giustizia, dei beni culturali, dell'ambiente, della ricerca e della tutela del lavoro, prevedendo un piano straordinario di assunzioni che si tradurrà in realtà negli anni compresi dal 2019 Le do qualche numero: 6.150 unità di personale delle Forze di polizia; come diceva il ministro Salvini, 1.500 vigili del fuoco; 725 unità per l'amministrazione civile dell'interno; 50 per la carriera prefettizia; 3.000 amministrativi per gli uffici giudiziari, cui si aggiungono 600 magistrati ordinari e ulteriori unità di magistrati amministrativi; 1.000 unità per il Ministero per i beni e le attività culturali; 420 unità per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1.000 ricercatori presso le università; 1.000 ispettori del lavoro.

di euro e degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. Infine, c'è uno stanziamento di 200 milioni aggiuntivi per il finanziamento dei servizi di natura operativa delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco. Oltre quanto previsto nel disegno legge del bilancio, il Governo sta individuando le modalità attraverso cui assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria ed educativo-scolastica.

che sinceramente non serve a niente. Voglio capire come fate a spiegare a un poliziotto, a un carabiniere, a un vigile del fuoco o a qualcuno che lavora nel settore della difesa o della polizia

Ricordiamo che i nostri uomini delle Forze di polizia rischiano la vita ogni giorno. I cittadini ci chiedono sicurezza - e su quello siamo d'accordo - ma le nostre Forze di polizia chiedono più risorse sia umane che economiche.

video. Il problema non è il video girato, anche se sarebbe vietato. Il problema è che in quel video mi si dà del pazzo e del fuori di testa. Può non piacere o essere mal considerato, magari da animi tracotanti,

ogni volta che entro in questa Aula, anche se sono alla seconda legislatura, mi emoziono. Sapere di dover intervenire per conto del popolo italiano e avere la possibilità di parlare

c'è la grande responsabilità di fare bene e di fare bene per quel che si sa fare, e facendolo al meglio. In conclusione, voglio semplicemente dire che sono fatto in questo modo. Cerco di fare bene il mio lavoro e, per fare bene, a volte ho bisogno anche di leggere, rileggere, correggere, ricorreggere. E, quindi, già vi dico che mi succederà ancora.

Signor Presidente, sarò rapidissimo. Come sa la Presidenza, quest'Aula lavora per una somma di effetti, quelli prodotti dal Regolamento, ovviamente, e quelli prodotti dalla prassi. Io vorrei sottolineare che oggi, nell'ambito della prassi, è il caso di lasciare agli atti un passaggio, che penso possa essere utile per regolare i lavori delle nostre sedute di *question time* da qui a seguire. Il ministro Fontana ha legittimamente - e lo ha esplicitato attraverso le sue parole - risposto a un'interrogazione che, appunto per sua detta, non corrispondeva e non era formalmente attinente alle competenze previste dal suo Ministero. Quindi, è come se avesse detto a quest'Aula che si passa dalla stretta attinenza alla affinità,

Dicevo che c'era effettivamente un'affinità tra la questione posta dal senatore De Bertoldi e la competenza del ministro Fontana e c'era un'affinità rispetto alle varie dichiarazioni rese dal Ministro stesso su tali argomenti. Quindi prendo atto volentieri, aggiungo - del fatto che il tema dell'affinità possa rientrare nella modalità con cui interagiscono Governo e Parlamento. credo si debba da oggi tenere conto del fatto che, nel momento in cui anche i partiti di opposizione e in ogni caso tutti i Gruppi parlamentari vorranno, in ragione di una evidente affinità,

avuto e si è preso la facoltà di rispondere, proprio in ragione di affinità e senza una stretta attinenza alle proprie materie di competenza.

Sarà mia cura verificare se, al momento dell'accettazione dell'interrogazione, non dovessero essere gli Uffici a indirizzare eventualmente l'interrogazione al Ministro di riferimento più pertinente per la questione posta,